del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, 2.28, accantonato, risulta assorbito da precedenti votazioni e pertanto non sarà posto in votazione. Avverto altresì che la riformulazione proposta dal Governo all'ordine del giorno G5.103, anch'esso accantonato, è stata accettata dal senatore Cioffi. L'ordine del giorno risulta pertanto accolto. Riprendiamo ora l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 14, accantonati nella seduta antimeridiana di oggi.

attenzione, riguarda il fatto che nel testo attuale vengono escluse dalle agevolazioni fiscali le pompe di calore, con la motivazione che di altri sgravi fiscali. Vorrei ricordare qui due questioni: l'efficienza energetica garantita dalle pompe di calore è molto, molto elevata ed è maggiore del 50 per cento rispetto a quella delle caldaie tradizionali.

includere tra gli interventi che possono beneficiare delle agevolazioni anche la sostituzione da parte delle imprese della copertura in Eternit con impianti fotovoltaici*.(Brusìo)*.

in cui abbiamo ascoltato una decina di associazioni di imprenditori (audite poi anche esternamente), tutti i rappresentanti hanno sottolineato con forza che un provvedimento di soli sei mesi non è efficace e che è necessaria una stabilizzazione temporale.

per poi stabilizzarla al 45 per cento dopo la suddetta data. Ciò potrà avvenire solo se decideremo, così come ci consiglia l'Unione europea, di procedere alla tassazione ambientale, perché è dimostrato che è possibile e necessario spostare la tassazione sui danni all'ambiente detassando i comportamenti virtuosi e quindi il lavoro. [DI

L'emendamento 14.201 mira ad includere le spese per l'installazione di unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento all'interno delle misure di detrazione, di cui all'articolo 1, 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e ad includere ulteriormente nella platea delle installazioni anche quelle delle pompe di calore elettriche ad alta efficienza che utilizzino in regime di autoconsumo l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e/o da pannelli solari.

recepita nel provvedimento in esame. Appare interessante sottolineare che il binomio pompe di calore elettriche ed energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento si deve leggere nel fatto che le pompe di calore sono energivore poiché consumano energia non producendola;

parere non ostativo sull'emendamento 14.900, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del secondo periodo con il seguente: "Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico". Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 15.201 (testo 2), 15.900 e 17.0.8 (testo 2)».

14.3, 14.5, 14.200, 14.8,

il parere è conforme a quello dei relatori,

Perché escludere ogni altro intervento finalizzato al raggiungimento della massima classe di prestazione energetica, che invece è una delle finalità di questo provvedimento? Per me, come norma di chiusura ci starebbe tutta, comunque ci rimettiamo all'Aula

semplicità e franchezza al collega Consiglio, con il quale ho avuto la stessa discussione in Commissione, che, ovviamente, sul merito di questo emendamento, così come del precedente, siamo assolutamente favorevoli. Voglio però richiamare il fatto che la normativa generale che riguarda il rispetto del doveri verso il fisco, e quindi l'evasione dei tributi, così come l'elusione della normativa nel campo della sicurezza, automaticamente automaticamente comporta la decadenza da ogni beneficio, come in questo caso. Quindi, non si può ripetere una norma generale già prevista. Ovviamente, siamo sensibili sul tema, e quindi un ordine del giorno che recuperi il concetto e lo valorizzi all'attenzione di tutti noi è positivo; eviterei però di inserire in una norma di legge questioni già assolutamente assodate e previste nella normativa generale che riguarda il fisco o la sicurezza sui luoghi di lavoro. Eviterei quindi di fare demagogia per restare al merito delle questioni.

Credo che sia un impegno assolutamente troppo generico. Si tratta cioè di sanare una situazione che riguarda decine di migliaia di famiglie che vengono discriminate rispetto alla possibilità di vedere utilizzati gli incentivi per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico. Ritengo che

l'Agenzia delle entrate e che credo il Governo si debba impegnare a cambiare per consentire a tutti i cittadini di avere l'opportunità di fruire delle deroghe.

il parere positivo

È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

che non poteva essere procrastinata ulteriormente da parte dell'Italia. Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno infatti anticipato la normativa statale in oggetto, notificando i relativi provvedimenti alla Commissione europea. Le nostre normative sono addirittura più stringenti e assicurano in modo più rigoroso il rispetto degli obiettivi di tutela ambientale e di risparmio energetico imposti dall'ordinamento comunitario. È stato a questo punto per noi fondamentale che l'Aula del Senato abbia accolto il nostro emendamento e introdotto nel provvedimento una clausola di salvaguardia che tutela i decreti attuativi provinciali già emanati Grazie, un esempio di riferimento per tutti gli operatori nazionali. Riteniamo fondamentale, sia sotto il profilo dei costi economici che per gli aspetti di tutela ambientale, Grazie, la definizione di requisiti minimi in ordine alle prestazioni energetiche degli edifici e le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche ed è importante incentivare 1'utilizzo delle fonti rinnovabili. Non deve però essere sottaciuto che - almeno nell'immediato - i soggetti che procedono a nuove costruzioni o a ristrutturazioni importanti di immobili esistenti devono sopportare costi aggiuntivi, perché i risparmi dati dal minore consumo energetico si manifesteranno solo nel tempo.

che ha voluto favorire tali interventi a mezzo della proroga degli incentivi per il risanamento energetico, rendendoli ancor più appetibili con l'aumento della detrazione dal 55 per Lo stesso dicasi per la proroga degli incentivi per la ristrutturazione edilizia con la detrazione del 50 per cento. Ringraziamo il Governo per aver chiarito, accogliendo un nostro ordine del giorno, che i tetti di spesa per interventi sulle parti comuni

può quindi essere cumulata con l'analoga agevolazione per i lavori interni e, in caso di risanamento edilizio di un condominio, il proprietario può, per ogni unità immobiliare posseduta, far valere fiscalmente un importo massimo di 192.000 euro, e portare quindi a detrazione un importo di 96.000 euro spalmato su dieci anni. Salutiamo con favore anche il ripristino dell'agevolazione per le pompe di calore e per gli impianti di geotermia e l'estensione delle agevolazioni per l'acquisto di mobili, con l'inclusione dei grandi elettrodomestici a basso consumo energetico, che anche il nostro Gruppo aveva richiesto. Purtroppo la situazione critica della finanza pubblica non consente, allo stato, di stabilizzare queste misure; auspichiamo quindi che questo possa avvenire con la prossima legge di stabilità. Voglio anche sottolineare che a livello europeo non esistono incentivi di questo genere o che siano ad essi neppure paragonabili, persino in Germania, che in questo campo si è mossa da tempo puntando sulle energie rinnovabili e abbandonando il nucleare. Siamo quindi all'avanguardia in Europa attraverso tali misure incentivanti e siamo convinti che queste, nel loro complesso, consentiranno di raggiungere obiettivi ambiziosi e in ogni caso

dai sottosegretari Baretta e Vicari, e annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. *(GAL)*. Signora Presidente, il decreto al nostro esame sembra essere un atto dovuto oltre che di buon senso. Contiene infatti norme per il recepimento di una direttiva comunitaria approvata in sede europea ben tre anni fa. Voglio ricordare che il termine ultimo per il recepimento di tale direttiva avrebbe dovuto essere il 9 luglio 2012, cioè un anno fa; come al solito, siamo in ritardo e l'urgenza che giustifica il decreto è dettata dalla necessità di evitare un'eventuale procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. L'Europa in questo caso ci indirizza verso la promozione del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Se consideriamo che il settore dell'edilizia rappresenta almeno il 40 per cento del consumo totale dell'energia dell'Unione europea, diventa facile valutare quanto sia importante migliorare le prestazioni energetiche dei nostri edifici, soprattutto se si valuta che l'Italia in questo settore sconta un ritardo piuttosto importante rispetto al resto d'Europa. Questa direttiva rappresenta un importante obbiettivo, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20, ovvero la riduzione del 20 per cento del consumo energetico entro il 2020; a questo si aggiunga la riduzione dell'emissione di CO2 di almeno un terzo, dovuta ad impianti di riscaldamento vecchi e in alcuni casi obsoleti. Inoltre, l'efficienza energetica rappresenta certamente una soluzione anche per il miglioramento della sicurezza energetica

per l'efficientamento energetico rappresentano davvero uno stimolo anche per quelle aree, come il Mezzogiorno, che in passato hanno aderito in misura minore rispetto al Centro-Nord a queste misure di sconto fiscale. Il Meridione ha scontato sinora la presenza di molto nero in edilizia, superiore al resto d'Italia. Quindi, è anche questa una buona prassi. Pensiamo pertanto di essere fiduciosi sul fatto che ci sarà un avvio dei cantieri anche al Sud, dove ormai sta diventando patrimonio comune l'idea che una casa che è efficientata energeticamente può avere anche un valore immobiliare maggiore. Per tutti questi buoni motivi, ribadiamo quindi il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà al provvedimento in esame.

che ho posto anche durante la discussione e la votazione degli emendamenti. È chiaro che il decreto-legge nasce opportunamente, per fortuna, per superare il *gap* anche nel recepimento della direttiva europea e, quindi, per superare una procedura di infrazione che ci sta ad indicare quanto sia forte il ritardo del nostro Paese in questo campo.

Sappiamo quanto sia importante nelle politiche ambientali l'utilizzo dello strumento della fiscalità (in questo caso delle agevolazioni fiscali) e anche il mettere in campo una strumentazione che sappia incentivare i comportamenti virtuosi e - soprattutto - che ci faccia superare il *gap* di cui ho prima

la stessa IVA che lo Stato incassa per gli investimenti fatti va a coprire una parte sostanziosa delle detrazioni. Quindi, si mette in moto un meccanismo virtuoso per quanto riguarda l'economia e i posti di lavoro.

in questi anni, in un momento di crisi molto forte del settore edilizio, abbia fatto bene accentuare tutta la parte che riguarda l'intervento sulla riqualificazione e la messa in sicurezza, anche ai fini sismici, così come poi si è risolto con l'emendamento

e, per quanto riguarda i condomini, di un anno. Quindi, ritengo che, purtroppo, non ci siamo ancora su questo terreno. È stato importante - lo voglio ribadire, e riconosco

Sulla questione della somministrazione degli alimenti e delle bibite è vero che in base all'indicazione europea bisognava adeguarsi, ma noi avevamo in mano lo strumento per differenziare.

motivi, ripeto, molto a malincuore, perché su un decreto-legge in materia di efficienza energetica, anche tenendo conto di alcuni miglioramenti che ci sono stati, avremmo potuto esprimere un voto pienamente favorevole, il mio Gruppo non potrà

Ciò rende l'incontro di questa giornata particolarmente importante, vista la delicatezza dell'argomento trattato, che ci porta a dover constatare come si sia perduta un'ottima occasione per un'azione veramente incisiva a sostegno di un reale rilancio dell'economia del Paese.

gli articoli del testo originale, circa 300 sono gli emendamenti presentati, di cui 50 sono quelli a firma del Gruppo Lega Nord e Autonomie. Tali numeri, signora Presidente, dimostrano l'attenzione rivolta a questo importante

emendamenti, quindi, non si è potuto discutere neppure l'oggetto perché considerati privi della necessaria copertura finanziaria. Entrando nell'analisi del testo, il decreto-legge si pone un duplice scopo: da una parte, rimediare alla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e, dall'altra, rilanciare alcuni settori della nostra economia. Le proroghe al 31 dicembre 2013 delle detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed acquisto di mobili sono un segnale importante, ma sicuramente poco coraggioso. Le agevolazioni rappresentano di certo un valido strumento di supporto alle imprese, ma non possono essere la regola; ne sostengono la crescita e ne agevolano lo sviluppo innovativo, ma sono temporanee. La sola proroga non è sufficiente perché l'economia e le regole che la governano hanno bisogno di certezza e di stabilità: un intervento normativo che esaurisce in pochi mesi la sua spinta propulsiva non tiene conto di queste regole. Signora Presidente, il 23,6 per cento del sistema produttivo italiano è rappresentato da imprese artigianali. In questo settore, l'edilizia e il suo indotto rappresentano il 63,9 per cento. Tra il 2009 e il 2012 hanno chiuso circa 11.500 piccole imprese di costruzione. La seconda fase della crisi del 2012 è stata così pesante che anche il mercato delle riqualificazioni (su cui, tra l'altro, avevamo fatto affidamento) si è contratto nonostante gli incentivi. Anche il settore del mobile e dell'arredo conoscerà con questo decreto una fase di crescita positiva, che esaurirà purtroppo il suo effetto in soli sei mesi. un'occasione mancata per un settore che racchiude tante piccole e medie imprese della filiera del *made in Italy*, che vantano la produzione di prodotti di alta qualità per i quali il nostro Paese è conosciuto in tutto il mondo. Alla luce di ciò, ci si domanda quindi perché concedere una proroga dalla durata così esigua, ma soprattutto perché non affrontare la questione delle detrazioni in maniera strutturale, non ricorrendo a proroghe, ma improntando - e da subito - nuovi interventi normativi a carattere permanente. Ci si chiede poi se non sarebbe stato opportuno, ai reali fini di un rilancio del sistema produttivo, affrontare quello che è da tutti riconosciuto come il maggiore ostacolo non solo alla crescita, ma addirittura alla quotidiana sopravvivenza delle imprese: l'accesso al credito. Oggi infatti le imprese sono in crisi, oltre che per il calo della domanda, anche e soprattutto perché non hanno le risorse necessarie per creare investimenti e quindi dare occupazione. La sempre più stringente attenzione verso la tutela delle banche ha infatti progressivamente inciso sul rilascio di liquidità alle imprese, determinando un vero e proprio ristagno economico che sta compromettendo l'intero settore economico-industriale. Il capitale, paradossalmente, non è che manchi, ma rimane bloccato dai sistemi a garanzia degli istituti di credito. Ciò sta impedendo alle imprese di improntare nuovi investimenti a vantaggio della competitività e dell'occupazione. Quindi, meno soldi ad imprese e famiglie, meno domanda, meno occupazione: è un circolo vizioso che neanche il recente provvedimento a favore dell'occupazione può da solo interrompere. Signora Presidente, questo Paese con una mano dà e con l'altra toglie, e spesso il tolto è maggiore del dato.

per risparmiare e per far sì che lo Stato sia meno pesante serve un lavoraccio che nessuno ha voluto fare: nessuno ha voluto mettere le mani in tali questioni perché è lì che ci si sporca le mani! Noi questo lavoraccio lo abbiamo affrontato e continueremo a farlo, signora Presidente! La ricetta l'abbiamo consegnata ad un cuoco poco accorto. Federalismo, costi *standard,* riduzione della spesa pubblica: questa ricetta avrebbe messo a disposizione risorse che non sarebbero provenute da nuove tasse, ma da un efficientamento economico del Paese. Per finanziare questo provvedimento si è invece agito solo ed esclusivamente sulla leva fiscale.

Ben 24 scadenze fiscali e contributive saranno a carico delle imprese tra novembre e dicembre. A fine anno questa situazione produrrà effetti drammatici per i bilanci delle aziende, in particolar modo per quelle di aziende che costituiscono la colonna portante dell'economia di questo Paese. Le aziende, già in forte affanno per la cronica mancanza di liquidità, dovranno versare entro la fine dell'anno, tra imposte, tasse e contributi, tra i 10.000 e i 50.000 euro. In questo decreto-legge, poi, potevano esserci i presupposti per aumentare l'occupazione, sopratutto giovanile: anche in questo caso è evidente che, per le ragioni prima esplicitate, la partita occupazionale sarà fortemente limitata negli effetti. Tutte le questioni che sono state dibattute dal presidente Letta in Europa saranno banalizzate semplicemente perché nessuno nessuno assume dei giovani, anche se non si dovranno pagare i contributi, se non c'è la possibilità di far produrre l'azienda. L'Europa ha proposto l'ennesima strategia per il rilancio dell'occupazione, soprattutto giovanile, forse non rendendosi conto, però, di essere stata tra le prime cause del pauroso stallo occupazionale in cui non solo l'Italia, ma quasi tutti gli Stati membri si trovano oggi. Questi anni di ostinato europeismo hanno dimostrato come la fredda e sterile politica del rigore finanziario e della stabilità dei prezzi abbiano, in realtà, il solo scopo di tutelare le banche attraverso la creazione di un'Europa finanziaria e non politica, dove l'interesse economico è anteposto al benessere dei popoli che ne fanno parte. Se vuole sopravvivere a se stessa questa Europa deve profondamente rinnovarsi ripartendo dai cittadini che la compongono, i quali non la vedono più come un progetto nel quale riporre fiducia e speranze, bensì come un rigido controllore pronto ad imporre drastiche misure economiche che spesso non lasciano margine d'intervento alle singole economie nazionali. Sono proprio questi ultimi i temi a cui il Governo deve dare risposte: riforma del lavoro, cancellazione dell'IMU e congelamento dell'attuale aliquota IVA. Solo in questo modo sarà possibile infondere nei cittadini una nuova fiducia verso le istituzioni e l'operato della politica dando un segnale di incoraggiamento anche e soprattutto alle imprese,

il canone RAI le famiglie risponderanno: articolo 81! Non abbiamo la copertura finanziaria. Quando arriveranno le tasse scolastiche da pagare, le famiglie risponderanno: articolo 81! Non abbiamo la copertura finanziaria. Quando arriveranno i *ticket* sanitari da pagare, risponderanno: articolo 81! Non abbiamo la copertura finanziaria. Quando arriveranno l'IMU, la TARES e l'IVA alle nuove aziende o a quelle che pensano di mettersi in competizione sul mercato, loro risponderanno: non abbiamo la copertura finanziaria e, quindi, articolo 81! orientamento di voto favorevole a questo provvedimento, esortando al tempo stesso il Governo ad ascoltare maggiormente le richieste che provengono dai cittadini e a rispondere in modo concreto e trasparente alle loro esigenze. E spero non si appellino all'articolo 81!

Noi, come Scelta Civica, siamo contenti di quello che siamo riusciti a portare a casa insieme al Parlamento, però vorremmo impegnare il Governo a fare in modo che queste agevolazioni possano diventare una prassi, che possano diventare

è importante tener conto di queste detrazioni, perché esse servono a mantenere un patrimonio immobiliare che in Italia è eccellente, per alcuni versi. Non dobbiamo dimenticare infatti che noi abbiamo

potranno usufruire molto di questo decreto-legge. Sicuramente i tempi sono molto brevi. Dal momento in cui una famiglia deve fare i preventivi e deve chiedere le autorizzazioni, sicuramente ha poco tempo a disposizione per fare

quindi, il fatto di dare delle regole e di rimettere tutto in piedi in una nuova ottica, che deve portare il nostro Paese da una parte ad un risparmio e dall'altra ad una struttura una struttura imprenditoriale più vivace nell'economia, sicuramente è un ottimo risultato. Per quanto riguarda i mobili e gli elettrodomestici, penso che abbiamo dato un segnale importante a tutta a tutta la filiera del mobile, che - come sappiamo - sta soffrendo molto, alla filiera del *design*, che è molto importante per il nostro Paese, e sicuramente anche alla filiera degli elettrodomestici (del bianco), che era una delle filiere più importanti fino a quindici a quindici o vent'anni fa. In questo ambito dovremmo avere il coraggio di dire agli italiani che va acquistato il *made* *in* *Italy*, perché ogni volta che noi acquistiamo un prodotto italiano teniamo fermo un posto di lavoro e abbiamo un disoccupato in meno. un disoccupato in meno. Quindi, è importante rigenerare completamente tutta la filiera del *made in Italy*, che è una filiera rilevante; quella del mobile è una filiera che, come *design*, ci fa essere protagonisti in tutto il mondo.

con un margine diverso. Deve essere importante per le famiglie poter programmare e sapere che dalle loro tasse, da quello che contribuiscono a creare nel Paese in

almeno in questo caso, dobbiamo cercare, insieme al Governo, di trovare una soluzione perché non è giusto tale aumento. Invece, secondo me, è giusto l'aumento dell'IVA per tutti quei prodotti che vanno che vanno in automatico insieme alle varie testate e che non hanno nulla a che vedere con i testi scolastici, ma che molte volte vengono vengono messi sotto la voce "testo scolastico" quando non hanno nulla a che fare con questo. Quindi, è importante non ricaricare sui libri di testo, ma anche non far passare sotto questo discorso questioni che non c'entrano nulla con la scuola.

Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che abbiamo esaminato contiene importanti disposizioni per ridurre i consumi energetici nel settore edilizio, che rappresentano il 40 per cento del totale di energia consumata nell'Unione europea. La riduzione dei consumi energetici - ribadiamolo - costituisce una priorità nell'ambito degli obiettivi 20-20-20 in materia di efficienza energetica; priorità, quindi, giustamente sostenuta dal 2007 in Italia tramite questo meccanismo di detrazione, che nel solo anno fiscale 2011 ha permesso permesso di istruire 280.000 pratiche per investimenti complessivi superiori a 3 miliardi di euro. È un dato molto rilevante, capace di generare un risparmio energetico complessivo in energia superiore a 1.400 gigawatt/anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 305.000 tonnellate di anidride carbonica, che - ricordiamo - è generatrice dell'effetto serra. Per capire la portata di questi effetti evidenziamo che la diminuzione dei consumi energetici in termini economici, nel solo anno 2011, ha generato un risparmio diretto nella riduzione dei costi della bolletta energetica pari a 220 milioni di euro, quindi abbondantemente oltre gli effetti sperati nel cosiddetto decreto del fare, ottenuti tra l'altro aggravando gli oneri dei produttori di energia rinnovabile. Quindi, ribadisco: è un risparmio superiore a quello che il decreto del fare adesso consentirebbe. Il dato è ancora più interessante quando allarghiamo la valutazione sugli effetti positivi e sulle ricadute che questo provvedimento ha già prodotto nell'ambito sociale, riportando che questo ha permesso la creazione di oltre 50.000 posti di lavoro nel settore sanitario-energetico-ambientale, e con la riduzione delle emissioni in atmosfera. Vorrei ricordare un aspetto che non è stato evidenziato da nessun collega: la combustione del carbone produce molti inquinanti e in Europa i fumi emessi principalmente dalle ciminiere delle centrali elettriche a carbone

Questo dato è riportato in una ricerca condotta dall'Università di Stoccarda, per cui non è un dato ambientalista. Vorrei ricordare che questo provvedimento avrebbe comportato anche una notevole emersione delle attività economiche sommerse (il cosiddetto nero). Noi qui diamo per scontato che si faccia tutto regolarmente, ma sappiamo benissimo che non è così.

mancanza di discussione soprattutto relativamente al cuore degli emendamenti presentati, cioè l'allungamento temporale del beneficio sino al 2020. Il decreto infatti, come sappiamo, si limita a concedere tale beneficio solo sino alla fine di quest'anno, sei mesi, decisamente troppo poco sia per le famiglie sia per le aziende, che hanno la necessità di programmare gli interventi. Qui viviamo in un mondo separato, non ci rendiamo conto che le famiglie, e soprattutto le imprese, hanno bisogno di programmazione a lungo periodo.

associazioni produttive, esperti economici, ambientalisti e anche il settore bancario. Ebbene, tutte queste associazioni, nonostante la loro diversità di obiettivi e di interessi, si sono trovate unite sulla necessità di migliorare il decreto in esame chiedendo di dare stabilità al meccanismo di detrazione almeno fino al 2020. Voglio sottolineare che tutte le associazioni hanno lamentato con forza la mancanza di una seria politica di programmazione industriale.

infatti, che nessuna legge è buona se non mette i cittadini e le aziende in grado di usufruire di tale legge. In questo caso, trattandosi di interventi di una certa rilevanza, era necessario anche un appoggio finanziario

nell'esame del provvedimento, in cui credevamo di poter discutere su queste proposte confrontandoci in merito alle considerazioni raccolte, la Commissione ha proceduto nel suo *iter* senza alcun approfondimento, approfondimento, ovviamente necessario per trovare una sintesi efficace al fine di rendere la disposizione funzionale allo sviluppo economico. In Commissione avremmo voluto dibattere sopratutto su quanto emerso nel confronto con i rappresentanti del settore produttivo e imprenditoriale auditi, in particolare su come individuare soluzioni, anche in termini finanziari, per rendere stabile il meccanismo della detrazione fino al 2020 con un *decalage* della percentuale detrattiva, e su come determinare una maggiore funzionalità della sua applicazione inserendo uno strumento di facilitazione dell'accesso al credito per realizzare tali interventi. Invece, siamo stati costretti a ripresentare tutte le proposte nuovamente in Aula, forse nell'ingenuo tentativo di aprire un confronto, così come chiesto dalle parti interessate dal provvedimento,

Siamo sicuri che le proposte presentate sulla stabilità dell'ecobonus fino al 2020, oltre ad essere condivise con le parti interessate, i cittadini e il settore produttivo, in quanto l'applicazione precedente ha già salvato numerose imprese dal precipizio della crisi, avrebbero potuto agire da stimolo per un rilancio dello sviluppo economico, sociale e ambientale da cui l'Italia sarebbe potuta ripartire. In particolare, avrebbero determinato un beneficio diretto ai cittadini e alle famiglie che avrebbero impiegato al meglio gli oneri dell'imposizione fiscale, da sostenere ugualmente, per migliorare la qualità della vita nelle abitazioni e beneficiare di una riduzione dei costi energetici di almeno il 25-30 per cento. In definitiva, oggi abbiamo assistito alla perdita di una grande occasione una grande occasione per riattivare il mercato edile, che ha perso 350.000 posti di lavoro e che sta letteralmente boccheggiando. Se aveste votato positivamente per l'allungamento dell'efficacia del *bonus* del 65 per cento sino al 2020, avreste letteralmente salvato tale mercato e buona parte dell'Italia.

È una scusa inaccettabile, perché i cicli industriali ed economici virtuosi che si sarebbero generati avrebbero compensato ampiamente le spese *(Applausi dal Gruppo M5S)*, come hanno dimostrato le esperienze precedenti di ecobonus.

la realtà è che le *lobby* del carbone, del petrolio e del gas sono ancora fortissime e vogliono che si continui a consumare moltissimo per riscaldarci d'inverno, rinfrescarci d'estate per produrre l'elettricità di cui abbiamo bisogno giornalmente per far funzionare l'Italia. La realtà è che siamo in presenza di un Parlamento ancora fortemente influenzato da queste *lobby* che da trent'anni ci governano. Queste votazioni che escludono l'allungamento al 2020 sono pertanto una sconfitta per i cittadini e il sistema produttivo italiano. Intervenire oggi in questo modo, senza una visione strategica di prospettiva che ci porti almeno fino al 2020, rischia non solo di produrre scarsi effetti positivi senza vantaggi concreti,

Nonostante tutto quanto è stato esposto e con la triste certezza che saremo costretti in breve a riaprire un nuovo confronto su questi temi, dichiaro il nostro voto che è solo formalmente favorevole per non incorrere in procedure d'infrazione presso l'Unione europea.

adempie ad un obbligo europeo, contribuisce al risparmio energetico, migliora la situazione edilizia del nostro Paese e contribuisce allo sviluppo economico e al potenziamento di una filiera edilizia e impiantistica e di imprese industriali ed artigianali in cui l'Italia è assolutamente attrezzata e all'avanguardia. Il lavoro dei relatori delle Commissioni 5a, 6a e 10a, il lavoro dell'Assemblea ed il confronto con il Governo, rappresentato dai sottosegretari Vicari e Baretta, hanno migliorato il provvedimento. Si sono trovate soluzioni ad alcuni problemi, come ad esempio nel caso delle pompe di calore. Dispiace che una parte della copertura derivi dall'aumento dell'IVA sugli allegati ad alcuni prodotti editoriali. In alcuni casi si tratta di coperture non assolutamente certe, perché l'aumento dell'IVA porterà probabilmente ad una contrazione sensibile del mercato. In altri casi si tratta di un vero e proprio errore: mi riferisco all'aumento dell'IVA su supporti tecnologici e libri scolastici per l'infanzia, per l'istruzione professionale e per i non vedenti. Sottolineo a tal proposito l'importanza dell'ordine del giorno unanime dell'Aula del Senato ed auspico che il Governo trovi una soluzione nei modi che riterrà opportuni.

sia le imprese sia i cittadini. È anche vero che stabilire un termine al 2013 significa incentivare a sbrigarsi, a fare le cose rapidamente. Per questo motivo il Gruppo del PdL voterà con convinzione questo provvedimento. che venga accolto l'invito europeo a dotare il Paese di una legge organica che preveda un programma pluriennale di incentivi atto a realizzare una profonda ristrutturazione degli immobili nel nostro Paese, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità della vita dei cittadini che abitano questi immobili; tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio energetico; tenendo conto della necessità, anzi della indispensabilità di avviare una seria politica di prevenzione antisismica. antisismica. Questo provvedimento avrà un senso e una validità se sarà seguito da un provvedimento organico che sviluppi una prospettiva nell'ambito degli anni. Non credo ci sia nessuna ragione contro: credo che tutto il Parlamento sia sensibile a questo argomento. Si tratta di trovare le risorse e le modalità

incentivare attività (quella dell'edilizia, quella dell'impiantistica, quella di imprese industriali e artigiane capaci nel *made in Italy*) che rappresentano una forza per l'economia del nostro Paese. In attesa di un intervento organico mi auguro che questo provvedimento venga approvato rapidamente, mi auguro che questo disegno di legge venga applicata bene

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora rappresentante del Governo, intanto rivolgo un ringraziamento ai relatori e ai Presidenti delle Commissioni competenti per il lavoro svolto su un provvedimento complesso, atteso e che porta, come è stato già detto, un po' di ossigeno necessario al nostro sistema economico. Apprezziamo lo sforzo la disponibilità che è stata mostrata durante il dibattito parlamentare su alcune questioni che, in particolar modo anche i colleghi del gruppo del Partito Democratico, hanno voluto sollevare, sollevare, a partire dalla questione antisismica, accolta in un emendamento approvato oggi, così come le modifiche all'articolo 14, per quanto riguarda le caldaie e le pompe di calore. Comprendiamo alcuni limiti del provvedimento, altri lasciano anche a noi qualche dubbio, e ci accomuniamo alla sollecitazione al Governo perché

Il senso profondo del provvedimento, però, lo condividiamo, e convintamente. La sfida, infatti, è quella di fare dell'efficienza energetica uno dei punti qualificanti del nostro Paese. Si tratta di una scelta verso la quale è necessaria una omologazione verso l'alto, che può e deve consentire una riflessione sulla qualità delle costruzioni, la loro integrazione nel territorio, la messa in sicurezza di quest'ultimo. Per questo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, dichiaro il nostro sostegno al testo in esame, che sancisce la conversione in legge del decreto-legge

Relativamente alle norme per corrispondere ai criteri di efficienza energetica indicati dall'Europa in ambito edilizio, vorrei ricordare che nell'Unione europea gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo globale di energia. Si tratta di un settore in espansione, quindi con un consumo energetico destinato ad aumentare. La sua riduzione, con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, costituisce misura necessaria per ridurre la dipendenza energetica e l'emissione da gas serra. Il tema dell'efficienza energetica quindi, anche grazie al richiamo europeo, offre la possibilità di divenire un catalizzatore per quella crescita economica qualitativamente elevata di cui sempre più abbiamo necessità. Da un lato, infatti, gli incentivi possono rappresentare una spinta anticiclica in un contesto economico sempre più depressivo e, dall'altro, con la diffusione e la crescita di questo settore economico, è da considerare possibile un beneficio per il mercato del lavoro. Non si tratta, quindi, di produrre a tutti i costi, ma di produrre meglio. Da sempre l'Italia è capofila nella manifattura di alta qualità e su questa base si innesta il decreto-legge; su questa strada si deve, a nostro parere, insistere per il futuro investendo le risorse disponibili. Il decreto-legge disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici nuovi e di quelli sottoposti a importanti ristrutturazioni, decidendo che ogni cinque anni vengano rivisti; introduce nuove norme di definizione degli edifici ad energia quasi zero e la redazione di una politica di potenziamento degli stessi tramite l'attuazione di un piano d'azione nazionale. In particolare, fissa il termine del 31 dicembre 2020 affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano ad energia quasi zero, anticipandolo al 31 dicembre 2018 per gli edifici di nuova costruzione occupati e di proprietà di pubbliche amministrazioni. Con l'istituzione di un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici e con quella dello stesso a cui viene vincolata le vendita e la locazione degli immobili privati occupati dalla pubblica amministrazione si introducono importanti elementi di garanzia, di sicurezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini. È importante che con l'articolo 17 si sia operata una modifica del decreto legislativo n. 28 del marzo 2001 in merito ai requisiti richiesti ai sistemi di qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, disciplinandone il riconoscimento anche sulla base dell'esperienza professionale, evitando così, nell'attuale fase di crisi economica, di negare a migliaia di lavoratori - artigiani, dipendenti o o titolari d'impresa attualmente in attività - la possibilità di qualificarsi e di continuare a operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora possibilità di crescita. Non possiamo, inoltre, non sottolineare l'importanza del potenziamento e della proroga del regime di detrazione fiscale introdotto con l'articolo 14 e con le modifiche a cui mi richiamavo poc'anzi, innalzando la detrazione al 65 per cento e prorogandola fino al termine di quest'anno; ciò consentirà innanzitutto di realizzare un risparmio di energia. I consumi civili rappresentano il nostro impatto più diretto.

con un taglio di emissioni di CO2 pari a 305 chilotonnellate. Sempre nel 2011, le richieste di intervento sono state circa 300.000, per investimenti superiori a 3.300 milioni di euro, con un valore complessivo degli importi portati in detrazione pari a oltre 1.800 milioni. Dai risultati citati nella relazione si evince il successo di questa formula,

L'aver prorogato il termine del beneficio fino a giugno 2014 relativamente agli interventi sui condomini, il cui consumo energetico è superiore alla media italiana già piuttosto elevata, consentirà una riqualificazione di intere aree urbane oggi fulcro dell'organizzazione sociale e civile delle nostre comunità. La spinta agli interventi di ristrutturazione edilizia potenziata con la proroga al 31 dicembre, l'innalzamento al 50 per cento delle detrazioni IRPEF e il raddoppio del limite delle spese ammissibili vanno nella direzione di una riqualificazione urbana oltre che della dinamizzazione di un comparto - quello delle costruzioni - fondamentale per la ripresa economica del Paese, così come i provvedimenti per l'arredo legati alla ristrutturazione incentivano l'economia di comparti industriali attualmente in sofferenza. Un'ultima considerazione politica: una delle sfide principali per i Governi europei, a partire da quello italiano, è quella di combattere l'impennata della disoccupazione, che ha ormai toccato il nuovo massimo livello storico, con un dato del 12,2 per cento, con quella giovanile al 38,5. Come sostenuto dall'economista Federico Caffé, nessun male sociale può superare la frustrazione e la disgregazione che la disoccupazione arreca alle collettività umane. Per questo è compito del Governo e del Parlamento ricostruire la nostra azione attorno a questo perno. Questa riflessione, in particolare, scaturisce dall'attuale condizione in cui versano le politiche industriali nazionali, sempre più avviluppate intorno a questioni puntuali e ormai incapaci di azioni organiche, ma anche dalla consapevolezza che uno dei capisaldi su cui investire per una nuova stagione di esse sia rappresentato dalla cosiddetta *green economy*. Il Gruppo del Partito Democratico, in conclusione, sostiene questo provvedimento convintamente, considerandolo però un primo passo che fornisce nuovo carburante per imprese e famiglie in una fase economica e sociale difficilissima che richiede scelte nette e selettive per il prossimo futuro.

come ho già avuto modo di dichiarare in discussione generale, che ho preso particolarmente sul serio, poteva rappresentare un'occasione importante per rimodulare le iniziative volte non soltanto ad ottimizzare le misure orientate all'efficienza energetica, ma anche e soprattutto a recuperare le potenzialità economiche del Paese, in un momento notoriamente complesso, ma buona parte di queste potenzialità, a mio parere, si sono disperse nei meandri della discussione politica e delle non chiare dinamiche parlamentari. E qui mi fermo, perché i miracoli a cui abbiamo assistito su taluni emendamenti che partivano da un parere negativo *ex* articolo 81 della Costituzione e che poi sono stati accolti confermano proprio questo.

Tutto questo ha di fatto limitato la capacità di intervento del Parlamento su un provvedimento importante che, a mio avviso, poteva essere affrontato con maggiore lucidità, più apertura, maggiore lungimiranza, invece di essere relegato al gioco di equilibri politici o agli interessi delle realtà direttamente coinvolte (e mi assumo la responsabilità di ciò che dico). Ulteriore criticità va rintracciata nel discutibile ruolo avuto dalla Commissione bilancio e dal fin troppo facile bollino di onerosità che questa ha posto sulla maggioranza degli emendamenti presentati. Queste dinamiche invitano a riflettere: il provvedimento, per quanto si configuri come strategico e - ribadisco - utile, porta con sé però questi elementi che contribuiscono a ridurne l'efficacia e dinanzi ai quali non si può fare finta di nulla, colleghi. Ho ritenuto pertanto opportuno evidenziare la mia posizione di dissenso rispetto al mio Gruppo. Proprio per questa ragione dichiaro il mio voto di astensione (e lo dico a malincuore) al provvedimento in esame.

materia di soggiornanti di lungo periodo, di rifugiati e di persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L'articolo 7 reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva

L'articolo 10 reca la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso. L'articolo 11 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE.

che ha portato anche a mediazioni necessarie all'interno della Commissione: nessuna componente politica, a mio avviso, è stata mortificata. C'è stata una discussione civile ed equilibrata fra persone consapevoli di quel che dovevano fare e di quel che abbiamo fatto. Ci avviamo adesso a dover discutere di tutto questo. Speriamo che lo stesso equilibrio che la Commissione ha avuto nel fare quel lavoro non venga distrutto da discussioni, come o da pareri di vario tipo che possono essere anche meglio interpretati. La verità è che, al di là di tutto (il Ministro me ne potrà dare atto), abbiamo appreso da lei

anche un'organizzazione vera. Non so se in Europa ci stiamo perché siamo convinti - io lo sono -, o perché ci siamo. Fin quando non avremo un approccio completamente diverso, saremo perdenti. anni abbiamo avuto penalizzazioni incredibili nell'agricoltura, nella pesca e nei vari settori. Siamo alquanto approssimativi: c'è un puntare il dito contro tutti, ma le responsabilità sul non utilizzo dei fondi sono solo dei Governi, ci sono dei ritardi, spesso, delle stesse Regioni, delle Province (ieri) e dei Comuni? Anche le organizzazioni datoriali quale tipo di progettualità danno? Protestano sempre, ma sono scarse nella progettualità e nelle proposte. è una sfida vera quella che attende lei, il Governo e noi tutti. I primi passi sono fatti: la sfida vera è far convincere tutti che siamo in Europa e che ci sono doveri che con queste norme stiamo superando. Siamo all'interno del 3 per cento del PIL: siamo come l'Europa ci ha chiesto, anche in maniera dura. Con queste due norme e con le altre, se approvate, noi usciremo fuori da tutte le procedure di infrazione comunitaria. In una parola, signor Ministro, troveremo a poter stare a testa alta. L'Italia è a posto, anche se bisognerebbe riflettere sul perché di tante procedure di infrazione nei nostri confronti. L'Italia è a posto:

ho capito da quello che lei ha detto, e dovremmo capirlo tutti, anche se si è lontani e distratti e spesso si è legati più ad altre piccole cose come sono passate prima, alla quotidianità, non vedendo che l'Europa può essere il nostro guaio, ma può essere anche il nostro futuro, se sappiamo ben ben difenderci ed essere a posto. Così ci mettiamo a posto e potremo difenderci seriamente. Già una battaglia è iniziata, quella sull'occupazione dobbiamo farne altre. Credo che lei potrà recarsi a Bruxelles, a Strasburgo, in maniera diversa dopo che tutto questo sarà fatto con serietà. È un'altra Italia quella che si troveranno di fronte. La colpa è di chi ha governato, ma anche di chi ha fatto finta di non vedere per tanti anni. Abbiamo l'abitudine di puntare sempre il ditino, ma non è così: ognuno di noi deve guardare le proprie colpe. Questo è. Tutti insieme: può essere un'opportunità enorme. Credo che potremo alzare la voce, signor Ministro. Non dimentichiamo - l'Europa deve ricordarlo, anche a scapito della stessa Germania e della signora Merkel - che l'Italia paga prezzi per la solidarietà per la pace nel mondo che la Germania non paga, che altri Paesi europei non pagano. E fossero solo prezzi economico-finanziari! Il prezzo è, anche in termini di vite Abbiamo avuto decine di morti. Questa è una cosa che conta, perché l'Europa spesso c'è sugli scenari più atroci grazie all'Italia, che non è certo il Paese più ricco di questa Comunità. Queste cose vanno rivendicate. Non si tratta di battere i pugni sul tavolo. Non possiamo stare a vedere la Gran Bretagna dire: «Pongo il veto al bilancio»:o gni tanto dovremmo avere il coraggio di dirlo anche noi, ma non per essere pretestuosi. L'Italia c'è, è cofondatrice

Dobbiamo fare sul serio. Come è stato detto; dobbiamo fare gli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo questa volontà? Non solo noi qui, ma il popolo italiano è pronto a tutto questo? Sono passi seri. D'altronde, abbiamo tutti la consapevolezza che o si esce insieme, in Europa, o si muore tutti insieme. Né qualcuno può immaginare di salvarsi da solo perché, come qualcuno ha detto, tempo le guerre si combattevano in Europa con i carri armati, con i cannoni e con gli aerei: oggi si possono fare anche con la finanza e con la politica economica. Tocca a noi far capire a chi oggi è più potente degli altri che è un bene anche per loro, perché solitamente poi le guerre le perdono. Non vorrei che perdano anche queste, e noi abbiamo un ruolo importante come Italia. Abbiamo la nostra capacità, la nostra inventiva, ma dobbiamo avere anche la nostra consapevolezza. Questo ho appreso e questo spero. [**Presidenza del vice presidente

portato avanti dal presidente Chiti. Ognuno di noi per la responsabilità che gli appartiene ha cercato di fare il possibile; non avrà fatto il meglio, ma abbiamo cercato di fare il possibile, di essere coerenti con il Governo, e lo saremo. Gli saremo vicini. Ringraziamo il ministro Moavero che è stato sempre presente.

Il mio intervento è stato più in questo senso: tecnicamente ci arriveremo con il Bilancio, con il confronto con i colleghi, con la presenza del Ministro, che non finisco di ringraziare, perché è stato presente come non mai, come pochi: è la verità. Esprimo

Il relatore sul disegno di legge n. 588, senatore Cociancich, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, onorevole Ministro, il mio compito è quello di illustrare sinteticamente il disegno di legge n. che è chiamato «legge europea 2013» a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 234 del 2012. Ricordo che, fino all'anno scorso, la legge comunitaria riassumeva al suo interno sia la legge di delegazione europea (testé illustrata dal senatore Tarquinio), sia la legge europea. Quest'ultima si caratterizza per il fatto che tende ad introdurre nel nostro ordinamento con immediata efficacia quelle disposizioni che si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento interno agli obblighi che derivano all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea e per evitare l'applicazione di sanzioni che conseguono a procedure di infrazione. In questo caso, si tratta di sanare venti procedure di infrazione, risolvere undici casi EU Pilot (che sono procedure di infrazione anticipate, cioè annunci di infrazione) e dare attuazione a due decisioni della Commissione europea e a due regolamenti. È molto importante per il nostro Paese evitare l'irrogazione di queste sanzioni, che dal punto di vista pecuniario possono incidere in maniera molto severa, perché possono arrivare anche a diversi milioni di euro. Mi sembra

la lunghezza del provvedimento, non mi soffermerò su tutti gli articoli, ma cercherò di concentrare l'attenzione su quelli che hanno presentato, nel corso del dibattito in Commissione,

quella della fiscalità, quella del lavoro e della politica sociale, quella della sanità pubblica e quella dell'ambiente; vi è poi un ultimo Capo che reca altre disposizioni in generale. L'articolo 1 tratta del diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, con riguardo in particolare alla tutela del *partner* convivente. L'articolo 2 del disegno di legge è stato ritirato dal Governo.

consentendo una concorrenza e una libera circolazione anche di tutte le altre guide, sia nazionali sia straniere. A questo proposito è stato predisposto un emendamento che consente una sorta di individuazione di alcuni siti di particolare interesse storico, archeologico e culturale nei quali sia possibile mantenere la richiesta di una particolare autorizzazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica. L'articolo 4 concerne una disciplina sulle tutele per i viaggiatori che dovessero stipulare viaggi con agenzie di viaggio con le formule «tutto compreso». L'articolo 5 riguarda le società di avvocati stabiliti, cioè avvocati stranieri che intendono esercitare in Italia la professione legale. L'articolo 6 introduce delle norme in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza. L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di tassazione di aeromobili. L'articolo 9 riguarda i trasferimenti di denaro all'estero ed introduce dei vincoli in materia di trasferimento simili a quelli sull'antiriciclaggio. L'articolo 10 concerne la riscossione delle imposte comunali e la facoltà data ai Comuni di affidare la riscossione

L'articolo 11 disciplina l'orario di lavoro della gente di mare. L'articolo 12 disciplina questioni in materia di lavoratori a tempo determinato le soglie necessarie all'interno delle aziende per determinare i diritti dei lavoratori a tempo determinato. L'articolo 13 introduce una nuova disciplina in materia di diritto al sussidio per i nuclei familiari a basso reddito che siano anche composti da cittadini di Paesi terzi. L'articolo 14 tratta un altro di quegli argomenti di cui si è lungamente discusso in Commissione e riguarda

A questo proposito, è stato rilevato che le sanzioni che attualmente gravano sui produttori che non hanno adeguato le gabbie non sono

l'autorità, la competenza al Ministero della salute. L'articolo 16 riguarda i prodotti cosmetici ed attribuisce sempre al Ministero della salute la qualifica di autorità competente. L'articolo 17 riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari. L'articolo 18 riguarda, invece, le acque di balneazione transfrontaliere. L'articolo 19 inerisce alla gestione dei rischi da alluvione, e in particolar modo definisce cosa deve intendersi per alluvione, escludendo, per esempio, allagamenti accidentali. L'artico 20 riguarda la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, quindi delle cave. Anche su questo sono state avanzate numerose proposte di emendamento. L'artico 21 concerne una nuova disciplina relativa alle pile e agli accumulatori, quindi, le modalità con le quali questi rifiuti devono essere riciclati L'articolo 22 riguarda lo smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'articolo 23 concerne la valutazione di impatto ambientale. le risorse idriche superficiali e sotterranee. L'articolo 25 riguarda i danni ambientali, con la previsione di sostituire la riparazione primaria e complementare compensativa con un risarcimento pecuniario. L'articolo 26 è uno di quelli su cui si è maggiormente impegnata la Commissione, perché riguarda la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, in particolare il regime delle delle deroghe di prelievo a livello regionale. Su questo vi sono stati numerosi emendamenti, e la discussione è proseguita fino a pochi minuti prima dell'avvio di questa relazione.

del Governo era stato proposto per estendere la protezione dei disegni e dei modelli industriali, secondo un decreto‑legge del 2011 che applicava la normativa del diritto d'autore in luogo di quella dei diritti dei marchi e dei brevetti. La Commissione ha ritenuto di sopprimere questo

normativa che a suo tempo ha riconosciuto particolari benefici a coloro che sono stati vittime o sono stati danneggiati dalle calamità naturali, europea in qualche misura ha ritenuto essere in violazione della disciplina che impone un divieto agli aiuti di Stato alle imprese. Anche su questo c'è stato un lungo lavoro da parte della Commissione, che poi si è tradotto in un'articolazione in una maggiore definizione di quella che è la rilevanza comunitaria del concetto di concorrenza, che fa scattare la soglia di questi eventuali aiuti.

Anch'io colgo l'occasione, che mi è data da questa relazione, per ringraziare tutti i membri della Commissione, il Presidente, gli uffici e il Governo per lo spirito di fattiva collaborazione che ha ispirato il lavoro, e che spero possa essersi poi sintetizzato in una serie di modifiche, le più limitate possibili, proprio per evitare che da un lavoro di riscrittura delle norme potesse poi risultare un'ulteriore la nuova formulazione, che ovviamente tiene conto di tante esigenze espresse in questi ultimi giorni, sia compatibile con la disciplina europea, consenta all'Italia di evitare l'applicazione di queste sanzioni e, al tempo stesso, consenta di tener conto di situazioni che dal punto di vista sociale ed economico sono parse particolarmente meritevoli di tutela. PRESIDENTE.

affrontiamo la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con un doppio *deficit*. Da un lato c'è il fatto che ne parliamo nel mese di luglio, quando invece avremmo dovuto tenere questa relazione

vantaggio che deriva non solo dalla sua competenza, ma anche dal fatto di avere ricoperto lo stesso incarico nel precedente Governo. La relazione è articolata in tre

europea; il capitolo II passa in rassegna i principali sviluppi previsti nelle singole aree tematiche in cui si articola l'attività dell'Unione europea; le priorità in materia di adempimenti dell'Italia, la questione relativa ai processi di infrazione, che tanto ci debbono angustiare e tanto dovrebbero vederci impegnati nella risoluzione delle problematiche ad essi connesse.

In relazione all'integrazione fiscale, oltre a ribadire la necessità di dare piena attuazione al *Six pack*, al *Fiscal compact* e al *Two pack*, la relazione evoca l'idea di un bilancio proprio dell'area euro, che abbia capacità finanziaria autonoma, attraverso l'emissione di *bond* europei. Sul piano della legittimità democratica dei processi decisionali dell'Unione europea, la relazione condivide la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni a livello europeo, nonché l'urgenza di una piena attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali. La seconda parte del capitolo I è dedicata al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. la posizione negoziale italiana, fondata anzitutto sul principio secondo cui il bilancio dell'Unione europea va considerato non come un costo ma come un investimento, e che deve servire anzitutto per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa; al contempo, ricorda che l'Italia è il terzo contribuente netto in termini assoluti al bilancio dell'Unione europea (dopo la Germania e la Francia) e il primo contribuente in termini relativi, con un saldo negativo stabilizzato negli ultimi tre anni su una media di circa 4,2 miliardi di euro. Su queste basi l'Italia ha esercitato la sua azione negoziale. Ha ottenuto una riduzione del suo saldo netto negativo a una media di circa 3,8 miliardi di euro per il prossimo settennio, ma la sua posizione favorevole all'aumento complessivo del bilancio dell'Unione europea non ha trovato il consenso sufficiente Il capitolo II tratta delle singole politiche dell'Unione e delle relative priorità nazionali. Nell'ambito delle politiche concernenti il mercato interno e la competitività, con l'Atto per il Mercato Unico II la Commissione ha individuato quattro motori per la crescita, che sono: lo sviluppo di reti completamente integrate; la mobilità di lavoratori e imprese; lo sviluppo di un'economia digitale; il rafforzamento della coesione sociale e della fiducia dei consumatori. Nell'attuale fase economica, lo sviluppo del mercato unico non è più considerato solo una delle leve possibili a favore della crescita, ma il fattore principale per incoraggiare la ripresa economica e lo sviluppo. Con riferimento alla proposta di regolamento sulla semplificazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, si rileva con favore l'attenzione posta dalla relazione sulla questione del conferimento di delega di potere alla Commissione europea. In particolare, si auspica che le deleghe riguardino solo aspetti non essenziali dell'atto legislativo, come prescritto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e come più volte ribadito dal Senato, nell'ambito dell'esame degli atti legislativi europei in fase ascendente. Riguardo al settore dell'innovazione e dell'Agenda digitale, dopo la sentenza di rigetto della Corte di giustizia sul ricorso presentato da Italia e Spagna in merito alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una di una tutela brevettuale unitaria tra 25 Stati membri, si pone ora la questione politica se aderire o meno ai due regolamenti sul brevetto unico europeo. Il mercato unico digitale è considerato un obiettivo importante da perseguire, tenuto conto del suo notevole potenziale in termini di crescita economica. Nell'ambito della revisione del quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato, la Relazione si sofferma anche sul regolamento cosiddetto *de minimis*, affermando l'inopportunità di un allargamento eccessivo delle soglie di aiuti ammissibili, in quanto ciò rischierebbe di favorire i Paesi che dispongono di maggiori risorse finanziarie pubbliche. Favore viene, invece, espresso per gli sviluppi in materia di esenzione dal divieto per gli aiuti alla cultura, per quelli per le calamità naturali, per il capitale di rischio e per l'innovazione. In materia di migrazione e asilo, la relazione ribadisce l'importanza di sostenere l'adozione di misure volte ad assicurare un'adeguata assistenza tecnica e finanziaria agli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori, nonché di sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle agenzie europee, come l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e di proseguire i negoziati con i Paesi interessati, al fine di promuovere una gestione condivisa dai flussi migratori. Riguardo al settore della giustizia e affari interni, si segnala la proposta di regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Nel settore della giustizia penale, nei prossimi anni sarà prioritaria la messa in opera di una serie di iniziative volte a garantire una migliore e più uniforme protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea e un miglior coordinamento delle indagini transnazionali in materia. In tale contesto è prevista l'istituzione di una Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. È, inoltre, di grande interesse l'annunciata proposta di estendere il Sistema europeo di messa in rete dei casellari giudiziari, attualmente limitato ai soli cittadini degli Stati membri, anche ai cittadini dei Paesi terzi nei cui confronti un giudice di uno Stato membro abbia pronunciato una sentenza di condanna, attraverso la creazione di un apposito archivio centrale europeo. Per le azioni di sostegno alla mobilità degli studenti e alla mobilità professionale dei docenti, la relazione sottolinea la necessità di promuovere la conoscenza delle opportunità di mobilità internazionale degli studenti e degli insegnanti, nonché di superare i relativi ostacoli normativi e organizzativi. Per quanto riguarda il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per mancata attuazione o violazione del diritto europeo, la relazione ne evidenzia la significativa riduzione ottenuta nel 2012, quando si è passati dalle 136 del 2011 alle 99 del 31 dicembre 2012. Per la prima volta dopo oltre 15 anni l'Italia è riuscita a scendere al di sotto della soglia delle 100 procedure. Tuttavia, con la mancata entrata in vigore delle ultime due leggi comunitarie per il 2011 e il 2012, il numero delle procedure è tornato al di sopra di tale soglia. Con l'entrata in vigore della nuova legge, la n. 234 del 2012, il Governo ha presentato il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea per il 2013, grazie ai quali si auspica

i cittadini italiani. Per molti aspetti potremmo essere considerati cittadini di una regione europea più che di uno Stato sovrano, perché le materie che incidono sulla nostra vita quotidiana sono ormai innumerevoli. Mi auguro che dal dibattito che seguirà

La relazione è stata redatta in base a quanto prescritto dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, ed è articolata in quattro parti. La prima riguarda gli sviluppi del processo di integrazione europea; la seconda concerne la partecipazione dell'Italia alla realizzazione delle principali politiche settoriali; tratta della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione, compresi quindi i temi della formazione e comunicazione in materia europea e il coinvolgimento dei cittadini, su cui dirò qualcosa più avanti; ed ultima parte descrive le politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari e la loro utilizzazione, nonché i risultati dell'attività svolta. Entriamo nel merito dei contenuti. L'attività del 2012 è stata dominata dai temi economici e finanziari, con l'obiettivo di mantenere la stabilità dell'area euro e rendere operative le misure di *governance*. È evidente e sotto gli occhi di tutti che il particolare il particolare momento congiunturale e la crisi strutturale che stiamo attraversando, che affligge i Paesi europei, non ha tuttora consentito - è inutile negarlo - di produrre effetti visibili. Ad onor del vero, anche alla luce delle notizie che oggi vengono dal *premier* Letta circa l'incontro in Europa, dei passi in avanti ci sono stati, ma non ancora con gli effetti sperati. Su deciso impulso del Governo, l'impegno politico del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 in materia di crescita economica si è tradotto nel Patto per la crescita e l'occupazione, che articola in modo organico le misure di rilancio da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio. Per quanto riguarda il rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria, da parte italiana si è espresso il pieno sostegno a favore di un credibile ed ambizioso processo processo di riforma, assicurando anche il coinvolgimento del Parlamento europeo e dei singoli Parlamenti nazionali. Le prospettive di riforma dell'Unione economica e monetaria si articolano su quattro assi: definizione di un quadro integrato nel settore finanziario (la cosiddetta unione bancaria); nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio; integrazione delle politiche economiche; legittimità e controllo democratico del processo decisionale. Per quanto riguarda il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la posizione italiana al tavolo è stata da un lato quella di migliorare il saldo netto nazionale e dall'altro lato quella di avere un approccio globale, ispirato ai principi di uso efficiente delle risorse, della solidarietà e dell'equità.

migliorare il saldo netto secondo principi di solidarietà ed equità. Ciò significa riconoscere che esistono di fatto beni pubblici europei beni pubblici europei che possono essere protetti unicamente, o in maniera più efficiente, a livello di Unione europea, riconoscendo il loro essere beni pubblici. Nell'ambito della dimensione esterna dell'Unione, l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale è stato predominante, e l'esigenza è di parlare con una sola voce. A tale proposito, la risoluzione ONU sullo *status* rafforzato dell'Unione europea in senso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite è stato un risultato per il quale il Governo italiano si è battuto. In tema di allargamento, il Governo ha lavorato per garantire un adeguato riconoscimento dei progressi negoziali registrati dai Paesi candidati, in particolare per la Serbia, il Kosovo e il Montenegro. E tutti quanti abbiamo salutato l'ingresso della Croazia nell'Unione europea In tema di politiche europee di vicinato, in particolare con riguardo alla sponda Sud del Mediterraneo, l'Italia ha rimarcato la necessità di fornire risposte adeguate alle istanze espresse dai Paesi in cui si è verificata la cosiddetta primavera araba, dal punto di vista del sostegno politico ed economico, ma anche

sviluppo, come diceva il collega che mi ha preceduto, l'Italia è il terzo contribuente al bilancio dell'Unione europea e il quarto contribuente al fondo europeo di sviluppo. Ovviamente, da questo punto di vista l'iniziativa è specificatamente rivolta al raggiungimento di obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015, con un particolare *focus* sulla sfida storica rappresentata dalla primavera araba e sul nesso tra migrazione e sviluppo. L'Italia ha sostenuto molto l'azione dell'Alto rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi in materia commerciale. Sempre in materia commerciale, e considerate le specifiche caratteristiche del sistema produttivo e industriale italiano, allo scopo di tutelare le sue tante eccellenze, il Governo ha sostenuto con successo la necessità di pervenire ad accordi commerciali equilibrati, mutuamente vantaggiosi e ispirati al principio di reciprocità, che perseguano in maniera incisiva e contestuale sia gli interessi commerciali sia la tutela del sistema produttivo degli Stati membri. Quindi, non una chiusura e una tutela, ma anche la possibilità di sviluppo. il Governo si è impegnato perché venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sulla etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto *made in)*. In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha chiesto alla Commissione di valutare possibili soluzioni alternative e di fornire una analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale,

Nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune, tramite le proprie Forze armate l'Italia è risultata nel 2012 il quarto Paese ad aver contributo per la lotta alla pirateria. affari interni, l'Italia si è impegnata per le problematiche connesse all'immigrazione illegale, anche se, da questo punto di vista, dobbiamo riscontrare forti resistenze da parte degli Stati membri non direttamente coinvolti nella gestione delle frontiere esterne, soprattutto di quelle marittime dell'Unione europea. Nell'ambito delle politiche relative al mercato interno si è avviato un processo di revisione delle diverse discipline esistenti per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le regole del Trattato. In tema di proprietà intellettuale, per quanto concerne la creazione del brevetto europeo (di questo tema abbiamo parlato lungamente con il Ministro, e sono state poi anche fornite indicazioni). Italia e Spagna avevano presentato un ricorso alla Corte di giustizia sulla modalità di utilizzo della cooperazione rafforzata. Ma

la fascia di età minorile. Nel settore dell'istruzione si è lavorato per enfatizzare il ruolo dell'educazione come strumento della Strategia Europa 2020 e sull'esigenza di modernizzare l'istruzione superiore attraverso cinque direttive politiche, sulle quali autorità nazionali e istituti di istruzione superiore stanno lavorando e si confrontano. Così come per la cultura, dove si è lavorato molto per rendere il tema della diversità culturale e l'accesso alla cultura un tema predominante, anche attraverso la promozione di *partnership* creative. Nel settore del turismo, interessante è la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo, che si propone di aumentare la fiducia e la sicurezza dei consumatori nei prodotti turistici e di premiare gli sforzi dell'industria per offrire servizi di qualità. Sulla sanità i temi affrontati hanno riguardato non soltanto la libera circolazione

alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, rispetto cioè a come muoversi eventualmente in situazioni di questo tipo. In materia di tutela dei consumatori si segnala l'approvazione da parte del Consiglio,

mette a disposizione circa 80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 con l'obiettivo di raggiungere il 3 per cento del PIL entro il 2020 e di potenziare la competitività globale del sistema Europa. politiche ambientali ed energetiche è un altro dei settori molto importanti su cui si è lavorato e anche questo Parlamento sta ponendo una grande attenzione, per promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento di politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali ed economici, quindi non più a compartimenti stagni ma secondo un ragionamento più complesso che utilizza sostanzialmente tre pilastri di riferimento (obiettivi al 2020 emissioni al 2050, migliorare la legislazione ambientale e transizione verso un'economia verde), dando priorità al raggiungimento di un mercato unico dell'energia per riuscire quindi ad avere lo stesso trattamento tra regolazione di fonti rinnovabili e tradizionali. Mi avvio a concludere sul tema delle politiche di coesione, su cui c'è un grande

La Presidenza informa che le proposte di risoluzione sulle relazioni precedentemente illustrate potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale. È iscritto a parlare è il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

nelle modalità di recepire le direttive comunitarie e di risolvere anche le problematiche delle infrazioni, oltre all'analisi della relazione sulla partecipazione dell'Italia al

abbiamo modificato la legge n. 11, approvata nel 2005, quando il sottoscritto presiedeva la Commissione affari europei alla Camera, insieme al ministro Buttiglione e ad altri componenti importanti che oggi sono presenti in quest'Aula, abbiamo iniziato un processo di modernizzazione che è stato concluso appunto nella passata legislatura, con la nuova normativa che oggi attuiamo. Credo però che, più che guardare ai contenuti dei documenti al nostro esame, che per la gran parte sono condivisibili, sia necessario fare una valutazione sull'Europa, su quello che si può e si deve dire, non ritenendo l'Europa un dogma, e su quello che bisogna denunciare quando ci sono, per così dire, degli eccessi all'interno delle discussioni che riguardano istituzioni europee, perché sono criticabili. Io mi definisco "eurorealista", non "eurocritico": guardo a ciò che funziona, guardo a ciò che effettivamente è utile ai cittadini, ma mi riservo quella libertà di poter criticare quando le cose non funzionano.

condividere questo tipo di atteggiamento e dobbiamo denunciare questa sorta di abusi, ma a tutti i livelli, non solo a livello di Commissione europea, di Parlamento europeo, di Consiglio europeo, ma anche di quelle assemblee che hanno che hanno magari uno spirito parlamentare, ad esempio il Consiglio d'Europa, dove a volte pure si eccede. La settimana scorsa, ad esempio, qualcuno proponeva un rapporto per quanto riguarda l'Ungheria, e si pensava di aprire una fase di monitoraggio per un Paese dell'Unione solo perché un partito ha vinto con il 66 per cento dei seggi, grazie ad una legge elettorale che definiscono truffa, ma che è stata approvata dalla precedente maggioranza, che oggi è è opposizione. E quindi un'Europa che va ad incidere nella vita democratica dei Paesi membri non può essere accettata, qualsiasi istituzione democratica sia, anche quelle che sono espressioni dei Parlamenti nazionali, come nel caso del Consiglio d'Europa. In quella in altri rapporti in discussione la settimana scorsa, parlando ad esempio dell'omofobia, si diceva che non era possibile lanciare certi messaggi o comunque comunicare un certo tipo di informazione, anche all'interno dei luoghi di culto, magari condannando determinati atteggiamenti che certe religioni non condividono, come ad esempio la sodomia: e noi dovremmo, da cattolici, non poter più leggere nelle chiese le lettere di San Paolo, ad esempio. Credo che questa non sia la strada che dovrebbe essere seguita. Allo stesso modo, credo che all'interno delle istituzioni europee ci debba essere un po' più di solidarietà e di realismo e che si debbano guardare in faccia le problematiche svestendosi dell'appartenenza geografica. I colleghi del Nord Europa vengono ogni volta a dire che loro sono solidali per quanto accade magari sulle coste del nostro Paese, a Lampedusa o in altre realtà della Sicilia e della Calabria, nei confronti dei migranti, non accettano che qualcuno ponga l'attenzione, magari chiedendo di aprire una discussione, su quello che accade a Stoccolma, con le rivolte degli immigrati di seconda generazione, o su quello che accadeva a Malmö qualche Anche questi sono degli atteggiamenti che non favoriscono la crescita di una comunità europea, che però deve essere basata sui popoli, sui territori, su quelle realtà che veramente nella differenza possono fare grandi queste istituzioni e possono fare grande un continente, basandosi sul reciproco rispetto, sulla tutela delle specifiche identità, senza dire di essere migliori o peggiori di altri, ma cercando di capire che è proprio nella differenza che può esistere questa ricchezza culturale e storica I documenti al nostro esame sono a volte molto burocratici. Quanto poi al recepimento delle direttive, ci sono ancora degli eccessi per quanto riguarda direttive di dettaglio eccessivo, che potevano essere riviste nel loro impianto e magari anche per alcune parti non sottoposte alla nostra attenzione, anche se capisco la necessità di avere comunque degli indirizzi e delle normative omogenee in tutti i 27 (adesso 28) Paesi dell'Unione europea. Non dobbiamo però pensare che con le normative di dettaglio, ovvero quelle direttive che analizzano problemi che spesso possono essere risolti dai singoli Paesi,

per risolvere le questioni internazionali, ma che ci fosse - per fortuna - un sano confronto diplomatico e istituzionale. Quindi, se questa è la strada che si vuol percorrere, si sta sbagliando, perché l'Europa può essere protagonista solo se si occupa delle grandi tematiche. Per occuparsi delle grandi tematiche serve quel coraggio che oggi che oggi non riesco ancora a vedere nelle istituzioni europee, perché esse non sono elette dal popolo, perché non sono espressione di quella volontà popolare che invece dovrebbe essere un punto di riferimento per tutti noi. Parlare del Presidente della Commissione europea e pensare ad una sua elezione popolare significherebbe dargli la legittimità di proporre

Ci interessa molto il processo in atto in Europa per quanto riguarda la questione bancaria e la questione economica. Purtroppo, abbiamo sacrificato parecchi dei nostri interessi interessi diretti, come Paese, e spesso abbiamo anche sacrificato gli interessi della parte più produttiva del Paese a una serie di ragionamenti, che tornavano poco utili

credo poco, soprattutto quando non mi vengono spiegati nel dettaglio. Questa è dunque la linea che bisogna tenere quando nelle sedi europee si vanno a difendere gli interessi di coloro

maggiore vocazione del Paese - a realtà confinanti straniere. Questa non è dunque la strada da seguire. I documenti al nostro esame, le politiche in campo europeo devono sempre tenere in considerazione quello che diceva un professore

la crescita degli alberi è rigogliosa solo se la potatura avviene in modo corretto, se non è eccessiva, se non è fatta a caso, ma è studiata ed è chirurgica. Dovremmo ricordare queste parole semplici, spesso anche quando siamo in ambienti europei.

onorevoli senatrici e senatori, da quando siamo entrati in questo Senato, circa tre mesi fa, ci vengono sottoposti testi di legge che presentano il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità. Ciò non perché in passato sia mancata la competenza professionale per adottare i necessari provvedimenti che servono al Paese, ma per una diffusa incapacità - o svogliatezza - nel prendere delle decisioni impegnative da parte delle forze politiche. Abbiamo capito una cosa: anche il Parlamento italiano è affetto dal fenomeno dell'«arretrato cronico» e di quella generale immobilità che è pratica diffusa presso molti uffici della pubblica amministrazione. Il risultato di tale ignavia lo abbiamo oggi sotto gli occhi: pagine e pagine di direttive accumulate durante gli anni, che si trascinano di legislatura in legislatura, senza mai trovare recepimento, e che sono oggi in scadenza. Questo fiume di norme che ci è stato presentato da un giorno all'altro rischia oggi, di trasformarsi in una serie di procedure di infrazione corrispondenti a sanzioni economiche pesantissime per l'Italia. E di questo, coloro che sono rimasti nell'immobilismo per anni dovrebbero sentirsi responsabili. Scorrendo le direttive a cui il nostro Paese ancora non ha dato attuazione, sorgono spontanee due riflessioni. La prima ha un sapore amaro: se prima di entrare nelle istituzioni si avvertiva un senso di arretratezza rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, oggi tale sensazione diventa una triste certezza. Confrontando le dettagliate norme che ci vengono proposte dal legislatore europeo, con il nostro pasticciato ed arretrato sistema normativo, pieno di falle e lacune, emerge chiaramente che l'Italia si è trasformata, lentamente ma inesorabilmente, da Paese promotore e motore dell'Europa a Paese del terzo mondo. La seconda riflessione va invece fatta sulla natura delle norme: appare chiaro che alcune sono molto controverse e che non si ha avuto il coraggio di affrontare fino al termine finale per la loro criticità etica. Altre sono state invece rimandate continuamente a causa di piccoli e grandi conflitti d'interesse, onnipresenti in qualsiasi settore del nostro ordinamento. In particolare, con questo intervento desidero soffermarmi sulla direttiva n. 36 del 2011, scaduta il 4 aprile 2013, in materia di tratta di esseri umani. Essa stabilisce che venga istituito in Europa un reato unico al fine di regolamentare e punire in maniera omogenea l'odioso fenomeno di chi abusa, rapisce ed approfitta dei soggetti più deboli, al fine di sfruttarli. Tale norma definisce un elemento di novità nello sfruttamento della prostituzione minorile e delle posizioni di vulnerabilità dei soggetti deboli, con espresso riferimento allo sfruttamento di minori attraverso la minaccia, la violenza fisica o anche la promessa di denaro. Tale formulazione, probabilmente, sarebbe risultata indigesta per il Governo precedente, soprattutto per il qui non presente ex Presidente del Consiglio. Forse - ma solo forse - l'introduzione dei nuovi reati relativi alla tratta di esseri umani, caldeggiata dalla direttiva europea, avrebbe potuto influire sui capi di imputazione addebitati al povero e perseguitatissimo ex *Premier*, portandolo ad una sentenza di condanna ancor più grave. È stato quindi meglio, in questo caso, tralasciare il recepimento della direttiva n. 36 del 2011, ritenuta troppo «divisiva». Tra scuse ed impedimenti trasversali, questo Parlamento non ha avuto il tempo di ratificare queste norme. Inutile dire che l'attività parlamentare è stata anche rallentata da quei soggetti che avevano ben altro da fare piuttosto che contribuire all'*iter* normativo, visto che la loro presenza presso questo Senato, in passato come ancora oggi, rasenta lo zero assoluto. Di sicuro non si è sentita l'urgenza di recepire la direttiva n. 93 del 2011 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tali temi sono stati ritenuti secondari e non meritevoli di puntuale attuazione. Le nostre Camere, infatti, sono state troppo indaffarate a produrre ed emettere leggi *ad personam* ben più importanti: la salva Rete 4, la legge sul falso in bilancio, la legge Cirami, il lodo Maccanico, la ex Cirielli, i condoni, l'indulto, il lodo Alfano, la legge sul legittimo impedimento, la legge salva Previti. Ecco, questo è stato impegnato a fare il nostro Parlamento negli ultimi venti anni, con il consenso trasversale di tutte le forze politiche: un'istituzione ad uso e consumo personale, e temiamo non sia ancora finita. C'è bisogno di riportare le istituzioni alla loro funzione naturale al più presto e ritornare ad essere protagonisti del nostro futuro, e non spettatori impotenti che subiscono passivi i dettami europei, senza più ormai alcuna voce in capitolo.

seduta odierna. Le relazioni introduttive hanno esaustivamente illustrato il carattere del lavoro che abbiamo svolto in Commissione e l'importanza di questo provvedimento.

i quattro relatori, ma soprattutto i primi due, hanno affermato, di recepimento di direttive e di adeguamento. Questa è la prima parte del lavoro che abbiamo svolto, e credo sia importante sottolinearla, perché comunque rappresenta un punto indispensabile. Noi abbiamo bisogno - come è stato detto - di metterci a posto, di svolgere un'attività legislativa che non ci porti a finire in infrazione, che non ci metta sempre nella necessità di recuperare una condizione di adeguatezza alle norme europee. Credo che questo sia un punto di cui si sottovaluta l'importanza. Lo ha detto il Vice Presidente della Commissione sviluppando la sua relazione. Non è soltanto una questione burocratica: avere le norme che corrispondono ad altre norme. Qui la questione è anche di collocazione del nostro Paese all'interno del dibattito europeo. Questo voglio sottolinearlo. È difficile chiedere più Europa agli altri e noi siamo spesso portati a farlo - se non siamo a posto, se intanto non siamo più Europa anche noi. devo dire che i richiami che spesso il ministro Moavero ha fatto precisamente in questa discussione hanno trovato un'accoglienza, anche se non è semplice. Desidero sottolineare questo punto per dire che se vogliamo chiedere più Europa e vogliamo che l'Europa superi gli egoismi e gli individualismi dei vari Paesi è necessario che noi svolgiamo compiutamente un processo di integrazione. Questo mi sembra un principio semplice, ma che dobbiamo valorizzare perché ci porterà a presentarci meglio alle assise europee, anche perché dovremo

La seconda e ultima riflessione che voglio fare è che risistemando la politica europea, accogliendo le direttive e superando le procedure di infrazione abbiamo anche l'occasione di risistemare certe politiche nazionali, certe leggi del nostro Paese, e guardare meglio a certe situazioni, a certi settori o a particolari gruppi di imprese che

a individuare rapidamente soluzioni nuove. Diversamente, gli equilibri non terranno e la situazione in qualche modo transitoria che abbiamo determinato non reggerà. Ecco, volevo sottolineare vale a dire l'esigenza di cogliere l'occasione della messa a punto delle politiche europee anche per alcune indispensabili risistemazioni delle politiche nazionali, comprendendo che ciò ci chiederà impegni positivi in questo senso. Mi fermo qui, signor Presidente, con quest'ultima notazione. Penso sia stato un dibattito serrato, che ritroveremo in molti provvedimenti che verranno trattati dall'Assemblea

proprio ieri pomeriggio in Aula abbiamo ricordato una grande donna, Margherita Hack; a lei, nota anche per l'impegno speso in difesa degli esseri senzienti, mi sento di dedicare il lavoro che tutti insieme abbiamo portato avanti in 14a Commissione per porre limiti più stringenti alla vivisezione. Potremmo inoltre dire oggi che, approvando il disegno di legge di delegazione europea n. 587, così come integrata in Commissione dall'emendamento del relatore 9.0.11 stiamo agendo nello spinto della massima di Gandhi secondo la quale: «La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali». D'altro canto il nostro Paese, sottoscrivendo il Trattato di Lisbona, ne ha anche recepito l'articolo 13 che recita: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Come ricordava anche il professor Picozza dell'Università degli studi di Roma, il principio del benessere degli animali costituisce dunque un principio generale del diritto comunitario in quanto inserito nel Titolo II del Trattato (disposizioni di applicazione generale), al pari ad esempio di quello della tutela ambientale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Così si pone in linea gerarchica sovraordinaria per quanto riguarda le politiche comunitarie, incluse quella del mercato interno ed in particolare della libera circolazione delle merci, come pure in materia di ravvicinamento o armonizzazione delle disposizioni legislative nazionali in materia di ricerca, sviluppo, ed ambiente. Ciò comporta, in linea di principio, che le singole politiche sopra considerate e anche quelle espressamente ricordate nell'attuale articolo 12, devono operare un bilanciamento di valori con gli altri interessi considerati dalle politiche stesse, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Intervenendo dunque in merito all'articolo 12 dell'atto ora in esame, voglio confermare la nostra massima attenzione sui temi che riguardano la sperimentazione animale, sui quali peraltro abbiamo realizzato in Commissione importanti passi in avanti, sia con l'approvazione a larga maggioranza dell'emendamento 9.0.11 (testo 2), sia per i pareri favorevoli del Ministro della salute e del Ministro per gli affari europei, che mi sento di ringraziare particolarmente per l'impegno speso. Credo sia opportuno ricordare che le ragioni scientifiche dell'utilizzo degli animali in ambito sperimentale sono per molti oggetto di critica. L'efficacia di questa pratica è messa in discussione a partire dalle differenze genetiche esistenti tra individui che non appartengono alla stessa specie. Proprio queste diversità, infatti, impediscono di estendere con naturalezza e consequenzialità i risultati ottenuti su una particolare specie a quella umana. A puro titolo d'esempio voglio citare alcuni dati: il 92 per cento dei farmaci che hanno superato le prove sugli animali viene scartato con le prove cliniche sull'uomo; la percentuale di predittività dei *test* su animali per l'uomo è solo del 37-50 cento dei risultati ottenuti sui topi discorda da quelli ottenuti su una specie assai simile come quella dei ratti. Questi numeri potrebbero essere già sufficienti a testimoniare quanto la sperimentazione scientifica sugli animali possa essere inutile e fuorviante nei propri risultati. Disincentivare tale pratica a favore di metodi alternativi che non vedano l'impiego di animali è prima di tutto, quindi, un dovere che trova la sua ragione anche nella tutela della salute umana. Al problema della validità scientifica dei suoi metodi si affianca la questione etica che viene troppo spesso nascosta e che non può essere ignorata. La ricerca della conoscenza non è uno scopo che permette di giustificare qualsiasi azione; anzi, essa deve essere sottoposta alle ragioni etiche, libera dalla discriminazione arbitraria che permette a chi detiene il potere di dominare i più deboli. È interesse comune dunque dunque che l'Italia si faccia protagonista di un cambio di marcia che ci possa quindi orientare verso una più ampia diffusione dei metodi sostitutivi e che recepisca la pressante domanda dell'opinione pubblica che chiede maggiori tutele nei confronti degli animali. È certamente importante sottolineare che una recente ricerca dell'istituto ha rilevato che ben l'86 per cento degli italiani è contrario alla sperimentazione animale, in qualunque forma essa sia condotta. Così come credo sia importante ricordare che, a tutt'oggi, tale pratica in Italia coinvolge un milione di animali l'anno.

Signor Presidente, la settimana scorsa l'ex senatore Sergio De Gregorio ha chiesto al giudice per le udienze preliminari il patteggiamento per il reato di corruzione nell'ambito del processo che lo vede imputato per la nota vicenda di compravendita dei parlamentari da parte del senatore Silvio Berlusconi,

ottenne 3 milioni di euro, 2 dei quali in nero, sia in contanti sia sotto forma di finanziamenti al suo movimento politico. Secondo le ipotesi di accusa quei soldi provenivano direttamente dal *leader* del Popolo della Libertà Silvio Berlusconi. De Gregorio in un intervista ha attribuito al senatore Verdini la seguente frase: «Dai Sergio, candidati! Andiamo tutti al Senato, io, te, Silvio, Nicola Cosentino. Ho visto i numeri, se ci facciamo eleggere, lì non c'è la maggioranza per far passare le ordinanze di custodia cautelare». Sabato 29 giugno Massimo Fini, riferendosi alle accuse della maggioranza al senatore Silvio Berlusconi basate su teoremi, ha spiegato la differenza fra un teorema e un assioma: il primo è una proposizione che trae delle conclusioni dandone una dimostrazione; il secondo è un principio che viene assunto come vero perché ritenuto evidente e non ha bisogno di essere dimostrato. La discussione in atto verte proprio sul fatto che esiste un assioma che dichiara Berlusconi innocente *ad interim* e appare indistruttibile. Qualcosa che può intaccare questo assioma si trova nella definizione di «patteggiamento» contenuta nel sito del Ministero della giustizia; si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino ad un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla scelta di questo rito speciale. Come Movimento 5 Stelle pensiamo che questa volta sia giunto il momento di prendere con la dovuta attenzione queste affermazioni, al fine di compiere un passo verso un Parlamento pulito e lontano da ogni sospetto.

non è un problema. Purtroppo in questi ultimi giorni ci sono stati due nuovi episodi. L'altro giorno, nella notte tra sabato e domenica, c'è stato un tentativo di incendio ad un mezzo di un'azienda che sta lavorando per il cantiere della TAV, opera probabilmente di frange No-TAV che si nascondono Questa mattina è stata recapitata - per fortuna è stata intercettata dai Carabinieri - all'ufficio postale di Sant'Antonio di Susa una busta con proiettili e minacce ad un imprenditore che ha lavorato, all'inizio della costruzione del cantiere, a Chiomonte e la cui unica responsabilità - com'è citato nel volantino e nella lettera allegata - era quella di aver collaborato con le forze dell'ordine

nella speranza di non doverne più fare, e per ricordare anche alla Presidenza, che se ne farà carico attraverso la comunicazione al Governo, che c'è ormai un pezzo, per quanto minoritario, che ha scambiato la Val di Susa

con l'obiettivo di farli rinunciare agli appalti regolarmente assegnati. In questo senso, nella giornata di ieri ho scritto che in Val di Susa siamo alla cultura di una mafia senza pizzo. La cosa non è ovviamente un fatto positivo.

difficilmente possiamo leggere, se non forse su qualche giornale indiano: ieri a Pinerolo un uomo è stato sbranato da tre tigri. Mi chiederete perché lo ricordo. Lo ricordo perché la senatrice Amati ha detto giustamente che Gandhi sosteneva che la civiltà di un popolo si vede da come vengono trattati e detenuti gli animali; ma io aggiungo anche da come vengono trattati gli umani che si occupano degli animali. Il sindaco di Pinerolo ha detto che quella era una morte annunciata, perché in questo Paese sono ancora troppi gli zoo privati, troppe le strutture che detengono animali esotici e selvatici in stato di cattività e sulle quali lo Stato fa finta di chiudere gli occhi. Finiscono così nella gestione esclusiva dei privati - immaginatevi cosa posso pensare io, da animalista, di un luogo di ergastolani innocenti, come sono gli animali chiusi nelle gabbie - e noi facciamo finta di nulla. Le tigri di Pinerolo si erano anche riprodotte; ci saranno cinque piccole tigri che per sempre saranno ergastolane

che si occupano di animali, così come sono troppi e abbandonati gli animali in cattività in questo Paese.